che dovrebbero occuparsi attivamente di questo problema, si attaccano al "Generale Inverno" con la speranza di frenare l'ondata di migranti invece di attuare politiche serie per la gestione e il governo di questo fenomeno. Alla luce di ciò, ci appare ormai chiaro che l'effetto macroscopico del salatissimo accordo tra Unione europea e Turchia sia stato quello di chiudere la rotta balcanica, facendo così scaricare sull'Italia e riguadagnare alla stessa il primato di Paese con il più alto numero di sbarchi di migranti irregolari. Dai *summit* di Ventotene, Bratislava e dall'ultimo Consiglio europeo è emerso chiaramente che l'attenzione delle istituzioni europee sui temi dell'immigrazione e delle frontiere esterne si concentra esclusivamente sui Balcani e sulla Turchia. Diciamolo francamente: l'Europa è sotto ricatto della Turchia, che ormai è un alleato inaffidabile che guarda con diffidenza, se non con ostilità, all'Unione europea, che intende ricattare

agli sfortunati che tentano di arrivare in Europa e a noi italiani che, in Europa, abbiamo l'obbligo di difendere le nostre frontiere. L'Europa guarda l'invasione in 27 modi diversi, si lamenta e si muove confusamente. I sogni europei sulla riallocazione per quote, sul *migration compact* e sul piano africano sono lettera morta. Non abbiamo notizie di nessun vero accordo. di ridistribuire l'onere dell'accoglienza e dell'integrazione, le istituzioni europee fanno la voce grossa ed impongono - solo a parole - a ogni Stato di fare la propria parte. Come rispondono gli altri Stati membri? Costruiscono muri o indicono *referendum*. L'Italia - che ha risposto diversamente - è stata lasciata con strutture di primissima accoglienza al collasso e, soprattutto, con un sistema per l'accoglienza di lunga durata inesistente, cosa che dovrebbe essere un problema di tutta l'Europa. Se siamo assolutamente incapaci di gestire l'accoglienza e l'integrazione di queste persone,

Per tamponare questa situazione, possiamo compromettere - questo è ciò che sta avvenendo - il sistema turistico sul territorio per dare una prima risposta a queste persone?

dove su quei barconi non arrivano solo disperati, ma anche molto terrorismo, che costituirà una minaccia per tutti noi. A pagare, di fronte all'opportunismo delle miopi politiche di questo Governo saranno solo gli italiani e quegli immigrati che le politiche sbagliate di questo Governo stanno trasformando da tragedia umanitaria a ricco *business* alimentato dalle vostre scelte miopi. Signor vice ministro Bubbico, avevate una opportunità stamattina

Dovevate farlo solo per questo: per dare più forza ad un Presidente del Consiglio che cerca di difendere gli interessi italiani in Europa. Oppure è solo uno *spot* elettorale? Oppure quella difesa antieuropeista messa in scena da Renzi vale solo fino al 4 dicembre? Noi ci auguriamo che valga anche dopo. Il Paese si deve ritrovare unito su questo. E quella mozione andava accolta, signor vice ministro Bubbico, proprio per lo spirito che poteva incarnare e rappresentare: l'unità di un Paese per difendersi da un grande attacco

che segue la risposta negativa alla nostra mozione da parte del rappresentante del Governo; un Governo che volta ancora le spalle ai sindaci, ai Comuni. Avevamo chiesto di rilasciare la carta di identità se non altro a chi ottiene uno *status* di rifugiato e di non concederla ad un semplice richiedente asilo, che le statistiche dimostrano che, per due terzi, risulta essere clandestino: richiesta bocciata. Abbiamo chiesto di imporre al gestore del centro di accoglienza di segnalare immediatamente l'irreperibilità del richiedente asilo

Abbiamo chiesto di non considerare, nella somma della popolazione residente - ai fini di impedire un incremento dei costi dei servizi in funzione associata

che una persona, un migrante ospitato nel centro di accoglienza, che quindi gode di vitto e alloggio gratis, possa incidere anche sui servizi di *welfare* comunali, visto che è assistito dallo Stato: il Governo vuole andare avanti così e allo stesso tempo non vuole ripristinare il reato di immigrazione clandestina, proseguire su una strada totalmente distante da quella della legalità e della deterrenza. È un Governo che pensa solo all'accoglienza. Non stupitevi, se gli sbarchi, da quando c'è Renzi, hanno raggiunto la cifra di quasi mezzo milione di persone; se quest'anno verrà superato il *record* del 2014, con 170.000 sbarchi. Non stupitevi se non siete in grado di gestire il sistema dell'accoglienza, che sta esplodendo. È di ieri il dato di 167.000 persone, di cui l'80 per

gli altri Paesi dell'Unione europea sono egoisti, quanto perché il Governo ha firmato un contratto che prevede il ricollocamento di persone con nazionalità

e troppo lenta è la giustizia ordinaria che spesso, come denunciano funzionari dello Stato, invertono il parere dato dalle commissioni territoriali. Dopo la bocciatura da parte della commissione territoriale, si trova un giudice che riconosce lo *status* di rifugiato per semplici

State perseguendo una politica scellerata che apre le porte soprattutto ai clandestini e scarica tutto sui cittadini italiani. Quest'anno

o, al massimo, di gestione di un'emergenza, senza un piano preciso per il futuro. Per quanto ormai la sensibilizzazione del Governo senza atti legislativi concreti non porti a risultati, intendo comunque votare a favore delle mozioni dell'opposizione. Appare chiaro che questo Governo dimostra di non volere o non essere capace di gestire l'emergenza migranti, causa anche il fatto che dobbiamo sottostare ai *Diktat* europei. Vediamo solo soluzioni estemporanee che ricadono sugli enti locali senza alcuna programmazione o l'affidamento al privato della gestione dell'accoglienza, alimentando così una economia distorta e a volte illecita, basata sul migrante come risorsa da sfruttare per finanziamenti pubblici. Appare evidente che accogliere persone a cui poi non si può garantire alcun futuro, se non di mero mantenimento in strutture sovrautilizzate, non è far loro Per questo devono venire in soccorso norme, come quella presentata da Alternativa per l'Italia, che regolamentino i flussi attraverso due precise istanze: regolare l'entrata dei migranti economici e preservare la dignità del migrante del migrante stesso spostando la linea di filtro fuori dall'Italia. Servono accordi per creare centri che permettano una formazione preventiva, informazioni sulla disponibilità di posti di lavoro

riteniamo che l'Italia stia facendo il suo dovere mentre l'Europa stia collezionando l'ennesimo fallimento perché è un'Europa impotente, schiava dei nuovi egoismi nazionali e incapace di far rispettare le sue stesse, innumerevoli direttive; altro che solidarietà! Credo, però, che nell'affrontare il tema drammatico contenuto nelle mozioni al nostro esame, oltre a tutto quello che è stato detto stamani, non si possa ignorare un altro dato ugualmente drammatico: quello che ci espongono i demografi. Si prevede che per mantenere sostanzialmente inalterata la popolazione italiana dai quindici ai sessantaquattro anni nel prossimo decennio, tenendo conto che gli italiani, sulla base delle dinamiche di fertilità e della speranza di vita, diminuiranno

È questo il fabbisogno di immigrati del nostro Paese. Volenti o nolenti questa è la realtà. Un numero necessario per compensare la riduzione della popolazione italiana in età lavorativa causata dalla diminuzione delle nascite e per salvaguardare l'attuale forza lavoro indispensabile per garantire la capacità produttiva e per rendere sostenibile lo stesso sistema previdenziale. Quindi gli immigrati sono attualmente un problema, ma saranno probabilmente una risorsa. Certo bisogna trovare un giusto equilibrio perché non si può mantenere l'immigrazione incontrollata. Ormai è stata superata la quota di arrivi del 2015 e si prevede anche il superamento della cifra del 2014, anno *record* per numero di stranieri approdati nel nostro Paese. Una situazione in cui l'Italia lamenta di essere stata lasciata sola da Bruxelles. A questo proposito, io credo che di fronte all'immobilismo dell'Unione europea, il Governo italiano abbia fatto la scelta giusta decidendo di inserire nella manovra proprio la spesa per la gestione dei profughi aprendo così, una volta per tutte, un contenzioso finale con Bruxelles. Un altro problema drammatico sono gli ormai 167.000 profughi accolti nei centri di accoglienza italiani ai quali si aggiungono 20.000 minori. Quello dei ragazzi giunti senza genitori o parenti è un problema drammatico. Quasi tutti vengono infatti tenuti in ostaggio dai trafficanti per costringere i genitori, spesso già sbarcati da noi, a pagare. Una vera e propria forma di ricatto. Questi ragazzi vanno inseriti in progetti educativi per sottrarli alla criminalità organizzata, invece più di metà di loro risulta dispersa sul territorio territorio italiano. Nella nostra mozione abbiamo sottolineato la necessità di un monitoraggio attentissimo dei centri di accoglienza straordinari, che accolgono il 70 per cento dei migranti, così come è indispensabile accorciare i tempi dell'esame delle richieste di asilo.

Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto «Alfano I» di Salerno. Benvenute e benvenuti al Senato.

esempio, che siamo di fronte ad un invasione, ma non c'è niente di più sbagliato e, se vogliamo vincere questa battaglia contro le falsità e contro l'assenza di cultura, per far crescere una logica dell'accoglienza, della comprensione e dell'integrazione, dobbiamo dare battaglia a questi luoghi comuni. Non c'è nessuna invasione, addirittura c'è la necessità, per il continente europeo, di valorizzare le tante migliaia di donne, di uomini e di giovani, che vengono spinti, in alcuni casi dalla disperazione e da dittature feroci e in altri casi da condizioni economiche disumane e da persecuzioni, a svolgere qui, in Europa e in Italia, lavori che non sarebbero assolutamente coperti dalle italiane e dagli italiani: penso ai lavori di cura nei confronti della persona,

di lavoratori extracomunitari, nelle nostre campagne italiane, vivono condizioni di completa e totale

a quello che oggi dipingiamo come un dramma, ma che può diventare un'opportunità storica nel processo di emancipazione mondiale dell'umanità.

le mozioni presentate oggi ci hanno consentito di aprire questo dibattito che evidenzia chiaramente dei concetti assolutamente contraddittori, come è chiaro che sia quando si parla di questi drammi umanitari.

l'Italia soffre particolarmente, più di ogni altro Stato europeo. L'Europa si trova al centro di un equilibrio tra le aspirazioni proprie dell'Unione di confermarsi area di pace,

emergenziale. In molte mozioni si è parlato di emergenza, ma io sarei cauto nell'utilizzo dei termini perché gli esperti ci dicono che questi flussi migratori persisteranno almeno per i prossimi venti

che sta applicando in maniera positiva delle misure importanti che ci hanno portato, rispetto a tre o quattro anni fa, ad una situazione migliore dal punto di vista dell'accoglienza. funzionano gli *hotspot*, funzionano la raccolta delle impronte digitali e l'identificazione dei migranti con il sistema Eurodac. C'è una convenzione con l'ANCI per una distribuzione più equa dei migranti

Si è parlato spesso in quest'Aula di *migration compact*. Su questo vorrei dire

negli Stati africani. L'idea è buona, ma come si fa a creare un ufficio laddove la gente scappa perché è terrorizzato in quanto priva della propria libertà?

Signora Presidente, lo scorso 3 ottobre si è celebrata la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Il 3 ottobre 2013 nel canale di Sicilia si consumò il più grave naufragio di migranti, costato la vita a 386 persone. Ma cosa è cambiato da quel giorno? Poco o nulla, da quello che possiamo vedere e da quello che abbiamo letto anche oggi. Ma soprattutto, quelle persone da cosa fuggono? fuggono? Fuggono dal Sudan di al-Bashir: due milioni tra morti e rifugiati; dal Congo di Kabila: sei milioni di morti; dallo Zimbawe di Mugabe, dal Sudafrica, dalla Guinea equatoriale. Fuggono, fuggono da posti che, comunque, noi europei

essere il modo migliore per permettere, sia ai Comuni che alle persone, di capire chi sono e da dove vengono i migranti e, in particolar modo, l'accoglienza dei minori stranieri.

Signora Presidente, il Gruppo di Forza Italia ha promosso, presentando una propria mozione, l'odierna discussione, il cui esito, anche se, ovviamente, non sarà da noi rappresenta un momento di chiarezza. Abbiamo presentato la mozione dopo che i Presidenti di tre Regioni - Toti della Liguria, Maroni della Lombardia e Zaia del Veneto - hanno redatto un documento che, con una decina di punti, ha sollecitato una politica più e severa nei confronti dell'immigrazione. Il Governo, attraverso i pareri espressi dal vice ministro Bubbico, è stato, nei confronti della nostra mozione, che riprende il contenuto di quel documento dei tre Presidenti,

Quanti soldi volete spendere, visto che dal 2011 abbiamo speso circa 12 miliardi? Quante sono le cooperative aderenti alla Lega delle cooperative che beneficiano di provvigioni di varia natura? Ricordiamo lo scandalo di Mafia Capitale e il ruolo decisivo di alcune coop rosse.

Quanta gente si pensa di ospitare? Badate che non c'è chi non condivida il discorso della solidarietà nei confronti di chi soffre. Sono 800 milioni le persone denutrite nel Sud del Pianeta e le persone in condizioni di povertà sono in più di un miliardo. Che facciamo? Le accogliamo tutte in Italia perché geograficamente siamo i più limitrofi? pure siamo per la solidarietà, ma l'Italia non può accogliere una quantità sterminata di persone. Perché in Spagna, vice ministro Bubbico, entrano 5.000 persone in un anno e in Italia abbiamo numeri spropositati? La Spagna dista dall'Africa 14 chilometri, nello Stretto di Gibilterra.

l'anno *record* degli sbarchi: siamo a oltre 166.000 arrivi, e solo più di 20.000 i minori. Abbiamo avuto, negli ultimi tre giorni, 12.000 arrivi. I terremotati che dobbiamo soccorrere nell'Italia centrale sono circa 4.000 e dobbiamo soccorrerli. Ogni giorno abbiamo un arrivo che equivale, supera o triplica il numero di italiani vittime del recente terremoto, ai quali pure dobbiamo dare una risposta. E lo accosto solo per far capire la gravità dei numeri, visto quanto per noi è grave e preoccupante la solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto.

Abbiamo anche un'altra domanda da farle: Forza Italia è favorevole al reato di immigrazione clandestina. Il vostro Governo ha avuto la delega, con il nostro voto contrario, per cancellare quel reato. Non avete esercitato la delega, per cui il reato c'è. Ma, siccome lo volete cancellare, pare che non ci sia più. Abbiate il coraggio di cancellarlo, così l'opinione pubblica potrà ancora di più condannare la vostra politica di resa nei confronti di questo fenomeno. Poi, se quel tipo di reato non va bene, studiamolo diversamente, ma in realtà voi avete la delega e non la esercitate, perché avete paura di cancellare il reato. E lo dico a quelli che invece condividono quella cancellazione. Chiedete al Governo che eserciti la delega contro la quale abbiamo votato, perché è un nostro

e ci auguriamo che il no degli italiani sia un no anche a una politica dissennata, che non è solidale, ma che sta solo esponendo l'Italia a una catastrofe umanitaria che ha poco di umanitario. della Marina militare, obbedendo a ordini dissennati del Governo - non siamo al soccorso di chi sta affogando, ma stiamo quasi andando a prendere i clandestini sulle spiagge per farli venire in Italia - poi viene pure processato per omissione di soccorso. Siamo solidali con la Marina per l'ingiusta accusa e anche per gli ordini sbagliati che Renzi le dà. Signora Presidente, le senatrici e i senatori del Gruppo Partito Democratico voteranno la mozione che ha come prima firmataria la senatrice Finocchiaro e sosterranno tutti gli impegni concreti e puntuali assunti dal Governo come sviluppo di un'azione incisiva Il tema delle migrazioni è oggi forse il più importante politicamente e culturalmente,

mette insieme politica economica, sociale e culturale e le rende politica a tutto tondo. Io penso che questo respiro non dobbiamo smarrire.

della senatrice Finocchiaro noi troviamo una visione seria e lungimirante: ci sono innanzitutto un respiro globale e la consapevolezza che le questioni hanno cause e soluzioni che non si riducono al nostro orticello di casa. Si parla di Africa, degli investimenti necessari per dare un futuro a quel continente; si parla di Mediterraneo, della cooperazione necessaria e della gestione dei flussi dei migranti. Il nostro Paese può e deve avere questo sguardo profondo, che è qualcosa di più della solidarietà: è parte della responsabilità di una Nazione C'è un'impostazione europea che abbiamo conquistato a fatica, anche facendoci sentire con forza negli scenari di Bruxelles, e che ora va attuata in modo compiuto. La revisione del Regolamento di Dublino, il *migration compact*, le nuove direttive per gli ingressi e i soggiorni per ragioni di lavoro, il piano di integrazione europeo che parla di scolarizzazione e solidarietà:

non solo salvare vite umane, che è la base di ogni civiltà - e io penso che non dovremmo dividerci su questo - ma anche lottare contro la migrazione irregolare e la tratta degli esseri umani, rafforzare e qualificare gli strumenti di accoglienza, perché anche questo è importante. In conclusione, noi incoraggiamo il Governo a proseguire e a rendere più visibili i nessi tra i vari interventi e a trasmettere un messaggio di forza e di saggezza, senza sottovalutare le paure, ma senza abdicare di fronte a esse, senza fomentarle per tornaconti di corto respiro. Se lei mi consente, signora Presidente, vorrei fare una riflessione finale sulla vicenda di Goro. Leggo su qualche sito di giornale una frase del tipo «A Goro vince la protesta». In tutta umiltà e con molto rispetto, credo

e diventa elemento per cui bisogna vincere contro qualcun altro e si fanno i blocchi per impedirlo, io dico che abbiamo perso tutti. Ha perso la politica, hanno perso le Forze dell'ordine, ha perso l'immagine del Paese e hanno perso anche quelli che credono di aver vinto, perché non è allontanando da sé l'onere di trovare soluzioni che si cresce. Anzi, si sono create nuove divisioni e fratture nella comunità e il circolo vizioso continua inesorabile. Più monta la paura, più si è fragili, e viceversa. L'impegno di oggi sia dunque un contributo anche a tutte le popolazioni, perché affrontino con forza e saggezza le prove che ci aspettano tutti. *(Applausi Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

su cui il parere del Governo è favorevole, in quanto accolte le proposte di riformulazione avanzate. Invito il senatore

Allegato B*). Passiamo alla votazione della mozione n. 663, su cui il parere del Governo è favorevole, previa riformulazione del quarto impegno ed espunzione delle lettere *b)* e *d)* del quinto impegno, oltre che del settimo e ottavo impegno.

numeri 1) e 3), lettera B), numeri 9), 10) e 12), nonché espunzione degli impegni di cui alla lettera A), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), e di cui alla lettera B), numeri 1), 6), 13) e 14).

essendo il nostro programma dei lavori continuamente sconvolto. Nel caso specifico, questa mattina la proposta del presidente Calderoli, fatta propria dalla Presidenza, si concludeva con questa votazione e non con il prosieguo delle altre mozioni, ma con gli altri punti già iscritti all'ordine del giorno. Su questo le chiedo veramente un minimo di linearità, altrimenti non riusciamo a organizzare i lavori del Gruppo, come succede anche agli altri Gruppi, in maniera decorosa.

Governo, colleghi, uno degli aspetti più controversi e dibattuti nell'ambito dell'impegno che viene profuso per il delicato, complesso processo di ammodernamento della nostra sanità riguarda il tema della continuità assistenziale. È un tema delicato, che viene affrontato non soltanto nelle sedi politiche dal decisore politico - in ambito legislativo nazionale e regionale - ma anche dalla comunità scientifica e da tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno competenza in questo ambito. Penso - per esempio - alle tantissime organizzazioni rappresentative dei pazienti affetti da talune patologie, prevalentemente di valenza cronica. Il tema della continuità assistenziale, dunque, assorbe in sé il principio di efficienza e di efficacia del servizio e di garanzia che il Servizio sanitario nazionale è nelle condizioni di poter dare al paziente, affetto da una determinata patologia, la sicurezza di una coerenza nel percorso terapeutico. E, quindi, si parla di continuità assistenziale richiamandosi spesso all'ospedale e al territorio, al territorio, con riferimento talvolta all'abitazione dove il paziente risiede, ovvero alle strutture sociosanitarie e assistenziali, per fare in modo che tutti i soggetti che a vario titolo operano - mi riferisco in modo particolare agli operatori della sanità - abbiano un codice per così dire unitario, linee guida unitarie a cui ispirarsi per dare principi di coerenza terapeutica. Un aspetto poco dibattuto, ma rilevante nell'ambito del tema della continuità assistenziale, è il delicatissimo problema di dare una risposta una risposta efficiente, efficace e appropriata a tutti quei bambini affetti da patologie che frequentano la scuola e che hanno bisogno, durante gli orari della loro permanenza negli istituti scolastici, di avere un'assistenza, in particolare nella somministrazione corretta dei farmaci. Il tema, per la verità, è poco conosciuto, ma gli addetti ai lavori hanno memoria di come e quanto il Governo e il Parlamento si siano cimentati per trovare risposte sempre più adeguate rispetto non solo

per la somministrazione di un farmaco, ma la competente e amorevole assistenza della maestra o del professore, i quali possono consapevolmente e responsabilmente svolgere una tale attività.

per una ricognizione dell'entità del fenomeno; per definire le linee guida, nonché il ruolo e la responsabilità delle figure professionali che andavano coinvolte nel percorso; nonché per definire una campagna di sensibilizzazione, formazione e informazione di tutti i soggetti. Al termine di un importante lavoro durato qualche anno, nel settembre 2015 sono state approvate le linee guida, definendo il modello organizzativo e procedurale per la continuità assistenziale terapeutica, con la condivisione dell'Autorità garante per l'infanzia con una consultazione che, su iniziativa di Federsanità, ha coinvolto tutto il personale docente. Le Regioni hanno espresso una valutazione positiva e, anzi, hanno sollecitato l'adozione dei provvedimenti di competenza. Giusto per dare un riferimento numerico, vorrei precisare che parliamo di oltre 45.000 bambini, di cui 20.000 affetti da diabete giovanile di tipo hanno naturalmente necessità di un'assistenza particolare. Accanto a loro ci sono anche i bambini affetti da asma ed epilessia. Stiamo parlando, quindi, di tre patologie particolarmente delicate che vanno affrontate

a sollecitare l'approvazione delle linee guida per la somministrazione dei farmaci a scuola, al fine di consentire il recepimento del lavoro che è stato svolto da una serie di professionalità competenti nella materia (mi riferisco non soltanto a quelle di estrazione scientifica, ma anche a

adeguare il sistema assistenziale durante il periodo di permanenza a scuola, soprattutto con riferimento alla patologia diabetica che, nel bimbo insulino-dipendente, necessita non soltanto della somministrazione dell'insulina, ma - mi si permetta - anche del sorriso rassicurante e premuroso

il Comitato paritetico svolga un'attività di vigilanza sull'attuazione del documento di indirizzo da parte delle Regioni e un monitoraggio finalizzato alla valutazione dei risultati che vengono ottenuti. Questo al fine di verificare che gli aspetti di ricaduta delle attività svolte in conformità alle linee guida possano rappresentare elementi di rassicurazione ovvero le eventuali criticità possano essere portate all'esame del competente Comitato paritetico per i necessari adeguamenti e le modifiche che si dovessero registrare. Questa è la

Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi per me è una giornata davvero particolare. Non sono qui in veste di senatore ma sono qui per raccontarvi le storie di centinaia, migliaia di padri e madri che, ogni giorno, lottano per garantire una vita serena e quanto più possibile normale ai loro figli. Le rinunce che queste persone sono costrette a sopportare per raggiungere tale obiettivo sono davvero infinite; molti, troppi aggiungerei, arrivano persino a lasciare il proprio impiego. Si autodefiniscono le mamme e i papà dei cortili perché tutti i giorni, per ore, attendono nei pressi della scuola dei figli, effettuando controlli periodici, intervenendo in caso di emergenza e provvedendo alla gestione dei pasti (pesano i carboidrati e valutando la quantità di cibo assunta dai bambini), così da somministrare la dose di insulina corretta. Tanta attenzione è necessaria perché in età evolutiva il diabete mellito è caratterizzato da una forte instabilità e, conseguentemente, da una gestione estremamente complessa a causa di peculiarità fisiologiche, psicologiche e nutrizionali che interferiscono in ogni aspetto della vita e delle esperienze del minore affetto da patologia diabetica e della sua famiglia. Molto è stato fatto in questi anni a livello nazionale e regionale per la gestione di questa insidiosa malattia - e colgo l'occasione per ringraziare la collega Granaiola e il collega D'Ambrosio Lettieri che da anni sono in prima linea su questo fronte molto è stato fatto, e mi riferisco in particolare alla legge n. 115 del 1987, al «Documento strategico di intervento per l'inserimento del bambino, adolescente e giovane con diabete in contesti scolastici ed educativi» e al «Piano sulla malattia diabetica». Ma troppi e troppo grandi sono ancora i problemi che i bambini e i ragazzi diabetici e le loro famiglie si trovano quotidianamente ad affrontare. Io oggi sono qui per loro, perché credo sia un preciso compito del Senato e del Governo, di tutti noi, alleviare il tremendo fardello che grava su queste persone e sui loro figli, un peso che per troppo tempo hanno portato in solitudine, magari facendo rete tra loro o con il supporto di un corpo docente che non esito a definire eroico ma dal quale pretendiamo forse troppo. infatti, che, pur nella necessità di formare dirigenti, insegnanti e personale ATA in merito alle malattie croniche, non possiamo pretendere che gestiscano terapie per patologie complesse e che richiedono la somministrazione di farmaci salvavita, come nel caso, appunto, del diabete. Infatti, come ricordato dal citato documento di AGD Italia, cito testualmente: «il diabete mellito di tipo 1 necessita obbligatoriamente la somministrazione di insulina più volte al giorno e si presenta con un quadro clinico di complessa gestione, sia perché investe tutte le attività basilari della vita quotidiana sia per la possibilità di scompenso dell'equilibrio metabolico che può mettere a rischio la vita stessa del paziente». Ecco perché ritengo sia ormai giunto il momento di superare un modello assistenziale incentrato sulla "volontarietà" degli insegnanti a somministrare agli alunni i farmaci in classe, a seguito di idonei corsi formativi. Sono insegnanti non infermieri! Non possono occuparsi anche della somministrazione di terapie così delicate, assumendosi responsabilità enormi che, in fondo, non gli competono, e non mi riferisco soltanto agli studenti diabetici ma anche agli asmatici, ai gravemente allergici o a quelli affetti da epilessia. Sono qui oggi perché spero che in un futuro prossimo non ci siano più bambini affetti da gravi patologie con difficoltà ad iscriversi presso asili, nidi e scuole, o che debbano rinunciare a gite e doposcuola; spero di veder sparire i genitori dai cortili e spero che questi genitori non siano più costretti a scelte drammatiche come mantenere il proprio impiego o prestare la necessaria assistenza ai propri bambini. È in questa direzione che la mozione a mia prima firma intende orientarsi, avendo, quale obiettivo generale, quello di garantire, in concreto, il diritto allo studio e alla salute di bambini e giovani affetti da patologia diabetica. Nel raggiungere tale scopo, si chiede non solo di dotare gli istituti scolastici nazionali dei mezzi necessari al fine di svolgere al meglio il loro ruolo nei confronti dello studente diabetico,

Si chiede, inoltre, la concreta realizzazione dell'obiettivo n. 9 del Piano nazionale sulla malattia diabetica, che sancisce la necessità di stabilire modalità organizzative, che consentano equità di accesso a microinfusori e altre tecnologie complesse (come i sensori per la misurazione continua della glicemia). L'obiettivo, quindi, è prevedere un rapido aggiornamento dell'elenco dei presidi per i diabetici. La mozione, infine, si sofferma sulla necessità di realizzare una revisione e un aggiornamento della normativa di riferimento, in modo da renderla organica, sistemica e rispondente alle esigenze emergenti. che la discussione delle mozioni che oggi ci troviamo ad esaminare costituisca un passo decisivo in questa direzione. Voglio credere che oggi cominciamo davvero a prendere sulle nostre spalle un po' del carico che grava ogni giorno su questi cittadini.

Che scuola è, se nessuno si prende la responsabilità di dare i farmaci? Che scuola è, se nessuno si prende la responsabilità di cambiare i ragazzi?

Che vita è questa? Chi li sta aiutando? Nessuno! Oggi sono molti i ragazzi - non solo Chiara - che non hanno i farmaci, molti non hanno l'insegnante di sostegno e viaggiano liberamente per i corridoi e molti non vengono cambiati, soprattutto al Sud. Mi rammarico molto, perché questi problemi non sono solo gravi, ma gravissimi e noi li trattiamo con una mozione, che presto si trasformerà in un'emozione e, poi, il nulla.

Per molti studenti si tratta di appuntamenti a cui non è possibile rinunciare, neanche nell'orario scolastico, sia per mantenere la continuità terapeutica, che per gestire i casi di emergenza. La scuola dovrebbe quindi provvedere a organizzare gli interventi necessari per assicurare alle famiglie la giusta assistenza, ma non sono pochi i problemi da risolvere; anzi, penso che siamo solo all'inizio di un lungo percorso. Mi piace citare alcuni esempi eclatanti, come quello di una bimba di undici anni a cui era stata diagnosticata l'epilessia, che per due anni non ha potuto frequentare la scuola primaria, nel suo istituto erano assenti assistenti per la somministrazione dei farmaci antiepilettici di cui aveva bisogno. Questo è uno dei casi eclatanti; nella maggior parte delle situazioni, fortunatamente, i bimbi e gli adolescenti affetti soprattutto da patologie croniche non vengono privati del loro diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione, ma il percorso che attende loro e soprattutto i loro familiari non è privo di ostacoli, anzi è spesso irto di grandi ostacoli. La somministrazione delle medicine necessarie alle cure e dei farmaci salvavita in orario scolastico è un problema quasi irrisolto, di cui si fanno carico soprattutto le famiglie, che diventano le uniche responsabili della cura. Alcuni genitori hanno addirittura rinunciato a lavorare per assistere il figlio e non privarlo di una vita il più possibile normale e di un percorso educativo e formativo che gli spetterebbe di diritto. È stata citata prima la costituzione del Comitato paritetico nazionale che ha dettato delle linee guida, ma oggi il vero problema è ancora quello di trovare chi somministra i farmaci. Se per la continuità terapeutica una famiglia può rapportarsi con la scuola, la prassi cambia di fronte all'emergenza; molte volte viene richiesta la procedura di urgenza: abbiamo citato il caso dell'epilessia,

di intervenire a livello normativo, per dare certezze che oggi non possono essere garantite. Ad oggi, inoltre, le linee guida regolano il problema in via del tutto generale, non entrando nello specifico dei farmaci da somministrare, delle relative patologie delle modalità di intervento, ma continuano a chiamare in causa i genitori, i medici di base, la scuola e soprattutto il dirigente scolastico. Ebbene, anche a questo riguardo molte volte il personale scolastico si è adoperato, ci sono delle raccomandazioni precise relativamente ai docenti e al personale ATA (come del resto per gli altri soggetti), che parlano di disponibilità e non di obbligo. quindi, delle raccomandazioni, ma il problema esiste, è importante ed è quasi ingravescente, tanto che anche l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha mostrato grande apprezzamento per l'attività del Comitato, sia per le modalità di lavoro, sia per l'utilizzo di importanti approfondimenti effettuati anche dall'ISTAT per quantificare e qualificare meglio il fenomeno. Allo stesso tempo anche l'Authority ci ha invitato a prestare attenzione ai diversi punti trattati, alcuni dei quali

bisognerebbe sempre immaginare un percorso capace di garantire l'appropriatezza del farmaco e dell'intervento in base alle varie situazioni, prevedendo la somministrazione di farmaci, non solo da parte di personale non sanitario, che deve essere adeguatamente formato, da parte di personale sanitario per i casi più complessi che necessitano di interventi differenziati. Sarebbe anche utile, signora Presidente, introdurre nel quadro normativo elementi temporali precisi, esempio il numero minimo di giorni che rendono obbligatoria per il dirigente scolastico la costituzione e convocazione di un gruppo di coordinamento. Inoltre, vista l'importanza di tenere sotto osservazione il fenomeno, si potrebbe anche rendere permanente e obbligatoria per tutte le scuole la rilevazione ISTAT; sarebbe altresì importante prevedere strumenti e modalità di valutazione e monitoraggio della corretta applicazione delle indicazioni nazionali a livello locale. Questo sta a significare che è un problema da attenzionare enormemente e sul quale sul quale tutti dobbiamo essere disponibili a portare il nostro contributo e a dare la possibilità al Governo di avere un quadro normativo di riferimento che possa dare finalmente soluzione al problema.

un Comitato paritetico nazionale, che studi proprio la somministrazione dei farmaci all'interno della scuola. Il problema è noto: non tutti i bambini hanno accesso alla scolarità, in quanto determinate patologie necessitano, purtroppo, di somministrazione di farmaci

I numeri destano preoccupazione. Più di 3.000 scuole hanno ricevuto richieste in tal senso e sembra che siano quasi 6.000 gli utenti, o le famiglie, che hanno espresso queste necessità

del personale scolastico, lasciando però alla volontarietà del corpo insegnante l'assunzione di questa nuova responsabilità.

del loro futuro ed è loro dovere. Ma ricordiamoci anche che questi farmaci hanno un costo e noi abbiamo una banda bassotti all'AIFA che non calmiera i costi.

*Pro domo* case farmaceutiche. Ovviamente ciò va contro il Servizio sanitario nazionale e il costo del farmaco nel Servizio sanitario nazionale.

risposte concrete e leggi conseguenti che diano aiuti a questi ragazzi e alle loro famiglie per far sì che possano avere una vita normale. Queste mozioni fanno riferimento alla patologia del diabete.

Signora Presidente, colleghi, siamo di fronte a un tema sicuramente importante,

per essere formato alla vita e che, a fronte di una patologia importante, magari abbia bisogno di avere un aiuto per la somministrazione di un farmaco per lui vitale. un genitore possa avere un momento di ansia rispetto a quanto credo sia un fatto assolutamente scontato ci deve far riflettere tutti. È qui l'importanza vera di questa mozione: farci capire

alla tematica che tale mozione porta alla nostra attenzione. Abbiamo tutti gli strumenti per poter essere iscritti a una società civile nella quale un bambino malato di malattie importanti, che

passo verso una civiltà completa nel nostro Paese sia un fatto normale e affinché in ogni scuola ci sia la possibilità di avere l'assistenza che il bambino merita. Non è un tema facile e non è un tema banale, perché siamo di fronte spesso anche a una incompetenza reale e non solamente di facciata: somministrare un farmaco è un'ansia e una grande

un salto di qualità alle nostre scuole. Tali linee guida sono state anche condivise dall'Autorità garante per l'infanzia e da Federsanità; le Regioni hanno auspicato un intervento in questo senso.

*(PD)*. Signora Presidente, voglio innanzitutto ringraziare i senatori D'Ambrosio Lettieri e Granaiola per questo lavoro, che è molto più importante di quel che si pensi, come abbiamo sentito dagli interventi. Di solito Di solito non si discute di simili aspetti perché si ritiene che debbano essere legati ai regolamenti. Però il problema - mi rivolgo alla Sottosegretaria - è terribile. Io ho ricevuto,

in ospedale; gli è stato dato un farmaco per bocca, ma i medici hanno detto che non andava bene. Ma non c'era nessuno che si sarebbe mai preso la responsabilità di curarlo. sarebbe mai preso la responsabilità di curarlo. Alla fine è arrivata una deliberazione del consiglio di classe, cui voglio leggere un piccolo pezzo, perché è sconvolgente, così almeno anche i colleghi hanno la percezione di cosa significhi: «I docenti e il dirigente ritengono che in questo momento da parte della scuola non sia possibile garantire la somministrazione del farmaco salvavita nei tempi e nelle modalità richieste dal protocollo. Si concorda pertanto che, non essendo possibile, nelle condizioni attuali, firmare un protocollo d'intesa per la somministrazione di un farmaco» - come se stessimo parlando della legge di stabilità, non di una persona e di un essere umano «in caso di emergenza si farà ricorso al pronto soccorso». Cioè, quando uno ha una crisi epilettica, notoriamente si telefona e si aspetta che arrivi il pronto soccorso; nel frattempo, hanno detto ai genitori del bambino di tenere un cuscino Questo è quanto. Ma quello che è peggio è che si dice: «Il consiglio di classe si rende disponibile ad attivare un progetto di scuola a domicilio, qualora la famiglia lo ritenesse preferibile ed opportuno». Vede, signora Sottosegretaria, io sono certa che lei inoltrerà al Ministro questa che non è una protesta, ma è l'espressione di una vergogna, in una scuola dell'obbligo dove il diritto alla salute viene negato. *(Applausi dal l'articolo 32 della Costituzione sia molto importante, ma è ancora più importante l'articolo 3, che parla dell'uguaglianza dei cittadini. In questo caso questo piccolo cittadino,

c'è un esempio emblematico di quanto l'Italia molto spesso si curi poco o niente dei suoi tesori e non trovi un modo per valorizzarli. A Coltano, una frazione di Pisa, si trova la storica palazzina in cui Marconi installò nel 1903 una stazione radiotelegrafica. I primi segnali inviati dalla stazione Marconi raggiunsero il Canada e l'Eritrea. Qui fu ricevuto l'SOS del Titanic e ottantacinque anni fa da questo luogo partì il segnale che illuminò il Cristo redentore di Rio de Janeiro. Nel corso della Seconda guerra mondiale, purtroppo, vennero distrutte sia le antenne che il fabbricato trasmettitori, lasciando però intatta la cosiddetta palazzina Marconi. Ebbene, questa importante testimonianza storica è oggi lasciata nel più completo degrado. Non è possibile che un luogo così straordinariamente importante sia abbandonato a se stesso. Si era parlato di un progetto per il recupero della struttura, che fu la più importante d'Europa per le trasmissioni radio continentali, ma tutto si è rivelato infondato e il progetto si è arenato. Ritengo sia di primaria importanza recuperarlo e restituirlo alla collettività. *(Applausi della

sempre che si abbia a cuore il patrimonio culturale e pertanto anche archeologico di tutti quanti noi italiani. di Punta Scifo, a pochissima distanza da Capo Colonna (zona sottoposta a vincolo archeologico), è esplosa una questione che ha avuto anche l'attenzione da parte del a seguito di alcune intercettazioni telefoniche riconducibili all'operazione "Aemilia", che appunto un paio di anni fa ha fatto comprendere che anche in Emilia-Romagna

mi piace definirlo con questo aggettivo - villaggio agrituristico a Punta Scifo potrebbe arrecare un danno, purtroppo irreversibile, a un patrimonio archeologico

per una questione che sta diventando esplosiva per la zona. Infatti, non si possono costruire 79 bungalow su base di cemento armato (per quanto poi vengano detti in legno), in una zona che, dal punto di vista ambientale, oltre che archeologico e pertanto culturale, merita solo rispetto. Giacché gli enti sono stati tra di loro contraddittori e giacché sono emerse intercettazioni telefoniche, a seguito di un processo penalmente rilevantissimo, come quello seguito all'operazione "Aemilia", chiediamo per l'ennesima volta al MIBACT, se c'è, di battere un colpo; altrimenti dobbiamo commissariare anche il Ministero di Franceschini.